mi auguro che i Gruppi ne tengano conto. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco dei contratti nel pubblico impiego. La mozione che ho presentato insieme ai colleghi Alicata, Fasano, Bernini, Fazzone, Malan, Piccoli e Aracri

intima al Governo di rinnovare i contratti. La mozione che illustro impegna il Governo ad applicare questa sentenza: può sembrare un fatto scontato, ma dall'estate dall'estate 2015 è passato un anno e mezzo e la sentenza non è stata applicata. La mozione discussa e approvata alla Camera l'11 ottobre era precedente alla presentazione della legge di stabilità

Intanto, lo stanziamento è per l'intero, rispettabilissimo, comparto del pubblico impiego, i cui contratti sono fermi da tempo, per colpa di tutti i Governi: questo lo dico io per primo, perché il blocco contrattuale si è trascinato in varie ere politiche.

a lei, come responsabile del Ministero dell'interno, per dire di metterci più soldi perché, pur rispettando tutto il pubblico impiego, la pubblica sicurezza, i Carabinieri e le altre forze di polizia vivono una condizione di disagio. Oggi leggo sui giornali, ad esempio, che un agente ferito a Firenze mentre difendeva una manifestazione promossa dal segretario del Partito Democratico (quindi dovrebbe stare a cuore a tutti il rischio che hanno corso quegli agenti) ha pagato il *ticket* all'ospedale.

punto *b)* si dice che si faranno delle assunzioni. Ben vengano le assunzioni. Lei sa, ministro Alfano, come ai tempi del Governo Letta il sottoscritto, con alcuni emendamenti, contribuì allo sblocco del *turnover* bloccato dal Governo Monti, però il *turnover* va ripristinato al 100 per cento e mi auguro che così avvenga.

questo cappotto di Napoleone, come si fa? Questo è il quesito aggiuntivo alla mozione ed è il lavoro ulteriore, ministro Alfano, che bisognerà fare alla Camera, mi auguro, e sennò al Senato, quando arriverà la legge di stabilità. Questi soldi devono servire per il contratto di tutto il pubblico impiego e del comparto sicurezza e difesa, per il riordino delle carriere e per confermare gli 80 euro. Lei ha detto più volte, anche in commissione al Senato, che farete il riordino del contratto e tutto Mi auguro che si faccia tutto. Questa mozione stimola il Governo a rispettare il lavoro delle forze di polizia. Non aggiungo altro, perché i minuti sono pochi ed è già mancato una volta il numero legale. La questione è chiara nella sua essenzialità e l'ho voluta affrontare senza calcare toni che potremmo facilmente calcare, rispetto al disagio delle forze di polizia e al loro sacrificio, che do per scontati in quest'Aula e ho citato l'episodio del *ticket*, che mi mi auguro che non sia vero, per dire quanto disagio queste donne e questi uomini stanno vivendo. Oggi il Senato ha la possibilità di mandare un segnale concreto di sostegno alle forze di polizia e alle Forze armate e anche una spinta al Governo per utilizzare la discussione sulla legge di stabilità in maniera positiva.

Salutiamo anche studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Cittadella -Margherita Hack» di Ancona.

parte dalla sentenza n. 178 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sospensione della contrattazione collettiva.

danni che sono stati prodotti non solo agli interessi legittimi di tutti i dipendenti pubblici,

Grazie

le vicende che hanno interessato drammaticamente il nostro Paese, dal terremoto di Amatrice a tutto quello che è accaduto e continua ad accadere nelle Marche e in Umbria, della necessità di rafforzare questo settore, in presenza di una situazione che vede

Questi sono i dati. Cosa era accaduto nella legge di stabilità per il 2016? I fondi che erano stati stanziati, compreso il contributo straordinario per le forze di polizia, per il Corpo nazionale

in modo molto chiaro di avviare tutte le iniziative per ottemperare alla sentenza rinnovando i contratti collettivi e soprattutto che nella legge di stabilità, con particolare riferimento ai comparti dei Vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, vi sia un'adeguata e congrua dotazione finanziaria,

i contratti e gli stipendi dei comparti dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle forze di polizia sono bloccati da oltre sei anni. Infatti, dal 2010, gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento ISTAT riguardo all'aumento del costo della vita. È utile ricordarlo quando parliamo di un settore della pubblica amministrazione così importante e delicato e oggi quanto mai strategico. Ciò nonostante, a oggi non risultano avviate trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze di polizia e delle Forze armate, costretti quindi a lavorare in condizioni di estremo disagio e con evidenti forme di illegittimità. Eppure, la Corte costituzionale si è espressa con grande chiarezza e ci auguriamo che quell'articolo 52, citato sia dalla senatrice De Petris che dal senatore Gasparri come la possibile soluzione almeno a una parte - a una gran parte, ci auguriamo noi - di questi problemi, sia davvero davvero approvato prima dalla Camera e poi dal Senato. Considerato che è stato recentemente avviato il riordino delle carriere delle forze di polizia a ordinamento civile, pensiamo sia importante

uomini e donne in divisa, evidenziando - casomai ve ne fosse bisogno - l'altruismo e l'efficienza delle forze di polizia, delle Forze armate e soprattutto del Corpo dei vigili del fuoco. Ma nonostante l'abnegazione di queste persone, continuiamo a non dedicare loro la giusta e meritata attenzione. Ecco perché riteniamo doveroso impegnare il Governo ad adottare tempestivamente iniziative per superare quella fase di blocco, avviando fin da subito le procedure negoziali per il rinnovo dei contratti, a stabilire lo stanziamento dei fondi per rilevare le cosiddette indennità accessorie dei poliziotti, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco che sono impegnati in servizi esterni, servizi che naturalmente aumentano il rischio per la vita e le loro responsabilità. Se fosse accertato che quel poliziotto impegnato negli scontri di Firenze abbia davvero dovuto pagarsi il *ticket* all'ospedale sarebbe una prova di grande inefficienza da parte di un Stato che, invece, deve avere a cuore innanzitutto la tutela e la protezione delle proprie forze di sicurezza. Noi chiediamo di introdurre a regime un sistema di tutela legale e sanitaria da parte dello Stato in in favore degli uomini in divisa, per assicurare loro le spese per i fatti inerenti al servizio, quindi qualcosa in più di quello che oggi già viene fatto. Chiediamo altresì che siano stanziati fondi per il soccorso pubblico, perché chiamare le forze di polizia e di sicurezza anche nei casi di calamità naturale vuol dire quantomeno dotarle di ciò che è necessario loro per svolgere questo servizio. Ci auguriamo quindi che la legge di stabilità sia l'occasione per riprendere un cammino di rispetto per quelle forze di polizia e sicurezza che, a dispetto della nostra disattenzione e nonostante il Governo non dedichi loro sufficienti risorse, continuano a svolgere meritoriamente il loro lavoro.

importante che venga affrontata oggi in prossimità della discussione del disegno di legge di bilancio, perché attraverso queste mozioni noi ci aspettiamo che il Governo e la maggioranza prendano atto dell'esistenza di un'emergenza che deve essere affrontata in modo efficace e dando risposte a una domanda reale del Paese. Come è stato detto dai colleghi, la richiesta principale è legata a un adeguamento delle retribuzioni delle Forze dell'ordine, cioè del comparto difesa, sicurezza e Vigili del fuoco. Questa richiesta non è volta a tutelare una categoria privilegiata, una richiesta sacrosanta che deriva dalla necessità di adeguare contratti - come è stato detto - scaduti ormai da troppo tempo. Ci si aspetta un rinnovo contrattuale su base

inadeguate a dare risposta a tutte le esigenze del Paese; bisogna però fare delle scelte in base alle priorità, alle emergenze e siccome la sicurezza in questo Paese è una vera e propria emergenza, ci devono essere risposte adeguate.

motivate, che abbiano un giusto riconoscimento del loro lavoro con organici e mezzi adeguati. Allo stato attuale questa circostanza non esiste nel nostro Paese. La scelta di questo Governo è stata quella di sopprimere centinaia di

voi avete scelto di effettuare tagli sulla sicurezza. Avete poi promosso un maldestro tentativo di introdurre il reato di tortura, quindi, invece di tutelare le nostre Forze dell'ordine, volete infierire nei confronti di coloro che compiono il loro dovere a tutela dei cittadini, è ormai all'ordine del giorno una serie di processi contro le Forze dell'ordine nello svolgimento del proprio mandato. Ad esempio, è di questi giorni la notizia di un carabiniere che ad Ancona, sparando per fermare un'auto che rischiava di

con una richiesta di risarcimento di 2,5 milioni di euro da parte dei parenti del deceduto: questo è il modo di tutelare la nostra sicurezza. Ci sono mezzi e materiali ormai obsoleti, agenti di polizia penitenziaria che si trovano in una situazione di grave disagio, disagio, vigili del fuoco che non hanno stipendi adeguati rispetto alle altre categorie e ai quali non vengono garantite prestazioni in caso di infortunio. A fronte di questa situazione drammatica, noi non vi chiediamo di tutelare queste categorie, ma di tutelare la sicurezza dei cittadini. Siamo convinti che le risorse che verranno investite in questo comparto, che chiaramente sono assolutamente

la seduta di oggi è inutile, non è vero che è utile. È una seduta inutile, come tutte le sedute inutili che abbiamo fatto negli ultimi tempi. In questa seduta discuteremo di una mozione

il Governo pronto a darne attuazione. Nessuna. È solo un esercizio per poter dire: io sono a favore, io sono contro; è solo un esercizio per poter

ai signori che ci stanno seguendo, dei sindacati di polizia, che sono qui presenti: andate a leggere tutte le mozioni: sono tutte pressoché identiche, perché ci mancherebbe che qualcuno non abbia a cuore il rinnovo dei contratti delle forze di sicurezza. Così come per tutte le mozioni

chi è che ha cominciato il blocco dei contratti della pubblica amministrazione? In quale Governo è iniziato il blocco? Vogliamo ricordarlo che era il Governo Berlusconi? Vogliamo ricordare che sono stati il ministro Alfano e anche il ministro Gasparri a farlo in quel Consiglio dei ministri? per la storia: non ero Ministro in quel Governo.

questa annosa situazione creata da loro e dai Governi successivi, che hanno continuato a perseverare in questo blocco degli stipendi di tutta la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle forze di pubblica sicurezza. E adesso il ministro Alfano ci verrà a raccontare, come è scritto nella mozione dalla maggioranza, che hanno stanziato quasi due miliardi di euro per il pubblico impiego: il Fondo nazionale per il pubblico impiego. Peccato che non ci dirà

come dal 2010 ad oggi, non arriverà niente, purtroppo, se non briciole!

Grazie con molteplici interventi, abbia disposto e reiterato la sospensione della contrattazione collettiva, la qual cosa ha comportato come conseguenza che le sigle sindacali più rappresentative non potessero sedersi al tavolo delle trattative per contrattare e ottenere nel comparto pubblico l'adeguamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali; la Corte costituzionale, con sentenza n.

le recenti emergenze sul fronte della sicurezza interna del Paese, e anche la minaccia terroristica sempre incombente obbligano

Nel tempo che mi rimane, ministro Alfano, vorrei puntare l'attenzione su un problema specifico, quello dei Vigili del fuoco. La medaglia d'oro che il presidente Mattarella ha annunciato di voler conferire alla bandiera dei Vigili del fuoco è un riconoscimento di altissimo significato simbolico e morale. Ora spetta al Governo e al Parlamento fare la propria parte. La legge di bilancio ha previsto dei provvedimenti in favore del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco, a cominciare dagli 80 euro strutturali da gennaio 2017 e dalle risorse stanziate per il rinnovo del contratto nazionale. Ora serve un ulteriore sforzo affinché i Vigili del fuoco non restino esclusi dal provvedimento finanziario per il riordino delle carriere previsto per il comparto sicurezza e difesa. Il personale dei corpi di polizia ed i militari avranno giustamente un finanziamento aggiuntivo, mentre per le modifiche dell'ordinamento del personale dei Vigili del fuoco non ci sarebbe, al momento, in previsione alcuna forma di finanziamento. Noi riteniamo indispensabile individuare anche per i Vigili del fuoco le risorse per questa fondamentale esigenza. Presidente, colleghi, ministro Alfano, non mi sembra inutile la discussione di questa mattina e lo dico perché non è un merito mio, né del Partito Democratico aver avviato questa discussione, che è stata invece avviata dalla mozione dell'onorevole Gasparri,

Grazie a tutti.

cattivo e spregevole - perché in sé è un fatto negativo - di una volontà politica particolare, ma essa è dovuta alla congiuntura economica che il Paese e l'Europa hanno vissuto. Certo, è cominciata col governo Berlusconi, ma è continuata anche oltre.

Devo dire, però, che già l'anno scorso c'era stato un piccolo stanziamento, che quest'anno viene sicuramente potenziato. Da parlamentare, e da prima firmataria della mozione della maggioranza (che abbiamo condiviso anche con tanti colleghi della maggioranza intesa in senso più ampio), devo

delle somme tra i punti *a)*, *b)* e *c)* e cioè quante risorse debbano essere dedicate alla contrattazione anziché agli altri impegni assunti con l'articolo 52, è un fatto che riguarda anche questo Parlamento. Quindi, la mozione impegna il Governo, ma impegna anche

per non fare soltanto l'inevitabile ma per fare tutto il possibile per dare risposte adeguate a categorie che da troppo tempo lavorano senza ottenere riscontri che meritano e che noi abbiamo il dovere di offrire.

tutto il comparto sicurezza e difesa sta testimoniando con una presenza veramente straordinaria. Ringrazio quindi il ministro Alfano e gli amici del comparto sicurezza e difesa.

Signor Presidente, ringrazio il Senato e in particolare modo i Gruppi parlamentari che si sono fatti promotori della discussione odierna. Ritengo sia una discussione tutt'altro che inutile, perché ripropone nel dibattito pubblico la questione della centralità delle Forze dell'ordine, della loro gratificazione, della collocazione del tema della sicurezza nell'ambito delle priorità del Governo. Sono certo che sia visibile a tutti come nell'ultimo triennio la sicurezza sia stata una priorità del Governo, non a chiacchiere, non a parole, ma con opere di bene, ossia con stanziamenti. Mi permetto, signor Presidente, di chiedere di allegare al mio intervento alcune tabelle che non sono tabelle di partito, ma sono venute fuori dai conti del Viminale, del dipartimento della pubblica sicurezza, che testimoniano

abbiamo fatto sì che, in un tempo di contrazione della spesa pubblica, la spesa in materia di sicurezza si espandesse, e lo abbiamo fatto in ogni ambito perché, se allegherò all'aumento degli investimenti per quanto riguarda anche le spese di funzionamento, le infrastrutture interne e tutto quanto attiene alla organizzazione, vi è un punto al quale siamo particolarmente affezionati, e cioè la valorizzazione del lavoro delle nostre Forze dell'ordine. Da quando siamo al Governo, nella sostanza abbiamo centrato alcuni obiettivi, che non voglio declinare per evitarvi un lungo elenco, ma ce n'è uno al quale siamo e sono particolarmente affezionato, che è lo sblocco del *turnover* che, superando un anglismo al quale non sono affezionato, significa che abbiamo ricominciato ad assumere lo stesso numero di persone rispetto a quelle che vanno in pensione. Prima funzionava diversamente; noi, in modo progressivo, abbiamo superato il blocco delle assunzioni e ora, nel 2016, sarà assunto lo stesso numero di donne e uomini delle Forze dell'ordine rispetto a quelli che nell'anno precedente sono andati in pensione. Questo è un dato oggettivo. Qual è l'obiettivo che ci riproponiamo in ambito legge di stabilità 2017 e anche anno solare 2017?

però noi lo centriamo con certezza. Siamo certi di fare un *poker* d'assi a favore delle forze di polizia. Voglio ripeterlo: stabilizzazione degli 80 euro, riordino delle carriere, rinnovo dei contratti e nuove assunzioni.

e sul tema del riordino delle carriere abbiamo stanziato le risorse necessarie e anche sufficienti. L'onorevole Gasparri, adesso nella veste di Presidente, faceva un riferimento ad un «ovvero» che avrebbe potuto rappresentare una condizione di alternatività tra la stabilizzazione degli 80 euro e il rinnovo dei contratti.

vi è un significato di un certo tipo, che giustifica l'interpretazione del presidente Gasparri, e vi è un altro significato che rimanda al concetto di «anche». Ora, non so quale dei due significati potesse avere in mente il funzionario del MEF che ha compilato materialmente la norma, ma a me compete l'interpretazione politica autentica, che è la seconda opzione del dizionario dell'Accademia della Crusca rinvenibile su Internet, e cioè la parola «anche». Noi faremo sia l'uno che l'altro: procederemo sia alla stabilizzazione del *bonus* degli 80 euro, che al riordino delle carriere.

i rappresentanti dei sindacati delle Forze dell'ordine per il rinnovo dei contratti e che le nuove assunzioni sono già in atto, per quanto riguarda lo sblocco del *turnover* di cui alle leggi precedenti, e le nuove assunzioni sono già finanziate con la legge di stabilità. Crimi sulla scarsa serietà di questa discussione. Infatti, quando si vuole negare un significato positivo si hanno molteplici argomenti per farlo e il senatore Crimi ha scelto quello di dire che questa discussione è semplicemente irrilevante. per parlare della rilevanza di questo nostro dibattito e ribadendo quello che in modo pertinente ha detto il presidente Gasparri

tale da consentire il piano di assunzioni straordinario, il riordino delle carriere e la stabilizzazione del *bonus* degli 80 euro, che pesa mediamente sulle retribuzioni per il 3,4 per cento. Cosa intendo dire con questa precisazione quantitativa?

i temi di cui stiamo parlando in questa sede vengono prima di tutti gli altri, per quanto ci riguarda. La prova sta nella circostanza che il ministro Madia si accinge a convocare i rappresentanti delle Forze dell'ordine proprio per affermare esattamente tutto questo e tradurlo dalle parole in fatti di Governo.

è una prova che non ha eguali in Europa o in altre parti del mondo. Vi faccio presente che il salvataggio non avviene in gruppo, ma una persona dopo l'altra e, quindi, solo la tempestività e l'efficacia dell'intervento hanno potuto consentire di salvare più

infatti finestre di assunzioni frequenti e anche numerose, al punto da poter dire che abbiamo incrementato la dotazione di circa il 10 per cento rispetto al totale dei componenti del Corpo nazionale Vigili del fuoco. Vi invito a considerare quale altra amministrazione pubblica o privata abbia incrementato il personale del 10 per cento in un tempo di contrazione della spesa. Questo si è potuto verificare per i Vigili del fuoco, a cui noi assicuriamo, unitamente alle altre forze di polizia, un incremento delle dotazioni dell'equipaggiamento e dell'infrastrutturazione interna (mi riferisco proprio alle dotazioni tecniche e ai mezzi che servono per la loro azione). Vi è un altro capitolo, più politico, che vorrei chiarire dal mio punto di vista perché aleggia nelle discussioni molto frequentemente, ed è quello dell'andamento della spesa e delle assunzioni in materia di sicurezza.

votante, consapevole di quel taglio e parte lesa relativamente alla polizia penitenziaria. Erano tempi di taglio della spesa ma le circostanze della politica e della vita, e anche una certa mia perseveranza, mi hanno dato la possibilità, che io ho colto con grande piacere, di rimediare a quei tagli, di rilanciare gli investimenti in materia di sicurezza e di rilanciare la politica sul personale delle Forze dell'ordine. Quindi sono vere entrambe le cose: c'è stato un periodo di tagli necessitati dalla crisi economica del drammatico periodo 2010 - 2011 e adesso che le cose vanno un po' meglio vi è l'affermazione politica della priorità delle Forze dell'ordine relativamente al tema della sicurezza che, a sua volta, è prioritario. Credo di avere detto, dal mio punto di vista, una parola di verità in questo ambito. Per quanto riguarda le mozioni,

Non torno indietro nel tempo, perché sarebbe inutile. Bisogna guardare ai fatti per quello che sono. Così prendo atto degli impegni che ci sono stati, totalmente insufficienti perché il momento è quello che è. Noi viviamo un dramma complessivo in questo Paese, subiamo purtroppo eventi sismici disastrosi, viviamo problemi di sicurezza generale che riguardano le forze di polizia e quant'altro incredibili. Ormai siamo alle rapine in autostrada ai pullman di passeggeri, non c'è più sicurezza, c'è la sensazione netta di uno Stato assente, specialmente al Sud - questo è un dato reale che è anche un limite alla crescita - e siamo ancora ai palliativi. Siamo in un momento di emergenza enorme, incredibile,

durante le manifestazioni e sembra che prima debbano morire e poi possano eventualmente difendersi. Non è possibile: su questo non si sente una parola, si continua a balbettare e a fare solamente politica,

nella legge di stabilità e cosa effettivamente si farà. Per ora lo riteniamo insufficiente non perché vi siano o no le risorse, ma perché in questo momento la priorità di questo Paese è: sicurezza, sicurezza, sicurezza. Questo è il dato reale da cui dipende quasi tutto. Non voler vedere questo e immaginare di fare *spot* elettorali è assolutamente ridicolo. Io non sono un tipo da pubblicità e resto decisamente esterrefatto. Per quanto riguarda la nostra mozione, il no proprio non lo capisco (forse perché c'è un riferimento alla magistratura). Qual è il no? Per quale motivo?

ciò è totalmente insufficiente per il momento che vive il Paese e per le risposte che vanno date alle nostre Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, che devono avere la certezza di essere non solo remunerati nel giusto modo per ciò che rischiano, ma anche tutelati nell'esercizio della loro funzione, perché questo spesso non accade. Ripeto che vengono massacrati e spesso anche incriminati; se è vero che quel poliziotto ha dovuto pagarsi anche il *ticket* all'ospedale, siamo alle comiche in questo Paese.

ma su questo non si dice una parola e ci sono solo palliativi. Qui servirebbero almeno altri 20.000 poliziotti: questo è il dato reale che dobbiamo affrontare. E ce ne usciamo invece con queste cose. Va bene così, noi continueremo la nostra battaglia, senza faziosità, solo vedendo i fatti. Semmai, ad aprile o a maggio le chiederemo

Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una situazione, quella che riguarda le forze di polizia, che è un qualcosa di assolutamente indecoroso e vergognoso per uno Stato civile. Ci troviamo in una situazione storica molto difficile:

e, non da ultimo, un problema come quello relativo alla retribuzione. Trovarsi con una sospensione dei rinnovi contrattuali da anni, che è stata sancita e dichiarata come illegittima sotto il profilo costituzionale, mette il Governo e la maggioranza di fronte ad una responsabilità enorme: una responsabilità enorme: quella di rimuovere ciò che è incostituzionale. Si deve quindi provvedere quanto prima a sistemare, rettificare e superare il blocco dei rinnovi contrattuali, in modo che gli agenti di polizia possano avere addirittura 150 euro in più in busta paga al mese. Al giorno d'oggi, nelle nostre condizioni, per una famiglia, per un agente, per una persona, 150 euro al mese significano tanto,

le Forze dell'ordine hanno dimostrato un grandissimo altruismo e una grandissima abnegazione, a prescindere da quei miseri salari che poi alla fine portano a casa ad ogni fine del mese, rischiando - come si vede dalle notizie di cronaca - non solo la propria salute,

assunzioni non servono assolutamente ad assicurare il ricambio necessario all'interno della Polizia di Stato. Alla fine, tenendo conto dei pensionamenti, l'integrazione, sebbene fatta, lascia comunque un grave scoperto di organico.

condividere con noi quello che abbiamo chiesto negli impegni della nostra mozione? Il rinnovo dei contratti, l'eliminazione della previsione della soppressione di 300 presidi di sicurezza sul territorio, il proseguimento del riordino delle carriere, le risorse per l'ammodernamento dei mezzi e degli equipaggiamenti,

Sentendo dire in quest'Aula che ci sono la stabilizzazione degli 80 euro, il riordino delle carriere, gli adeguamenti economici, lo

fa ritenere che, per la prima volta, un Governo abbia fatto il suo dovere. I colleghi che mi hanno preceduto hanno avuto la fortuna di essere rappresentati al Ministero dell'interno, ma interventi

Presidente, non chiederemo al Ministro la ragione per la quale invita il Senato a votare in modo schizofrenico (a votare a favore della stessa cosa e contro la stessa cosa nella medesima seduta) perché ne comprendiamo il motivo: una visione una visione un po' corta della politica e, soprattutto, del rispetto che si deve ai lavoratori pubblici, in modo particolare, a quelli delle Forze dell'ordine e delle Forze armate.

Proponiamo di avviare immediatamente iniziative per ottemperare a quanto è previsto dalla sentenza della Corte costituzionale. Badate che la Corte costituzionale interviene a rimuovere gli effetti di una decisione adottata a suo tempo da un Governo e da una maggioranza della quale faceva parte lo stesso ministro Alfano. Quindi, egli prima ha tolto e poi divide il Parlamento quando il Parlamento vuole restituire

incorrendo nella sanzione della Corte costituzionale anche in ragione del fatto che la sospensione della contrattazione si accompagna all'impossibilità

miglioramenti economici che sarebbero stati prodotti con la contrattazione collettiva regolarmente in funzione richiedono un esborso finanziario che oggi il Governo non è disponibile a fare; anzi, lei stesso Presidente ha detto le dotazioni finanziarie previste in legge di stabilità sono molto lontane, lontanissime dal poter coprire integralmente il danno già fatto. Pertanto voteremo a favore della nostra mozione, con cui chiediamo di destinare al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, con particolare riferimento ai comparti dei Vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, una dotazione finanziaria che sia significativamente destinata anche a colmare quel danno che purtroppo hanno creato una maggioranza di cui il Ministro faceva parte e un Governo di cui era sostenitore:

gravissimo che ha anche generato disaffezione e una lesione di tipo morale nei rapporti tra lo Stato, chi lo governa, e le Forze dell'ordine e le Forze armate che lo difendono.

signor Ministro, le mozioni oggi all'attenzione dell'Aula sono giustamente finalizzate a richiamare l'attenzione del Governo su una questione irrisolta.

la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, che ha sancito l'illegittimità costituzionale del quadro normativo su cui si è fondata la sospensione della contrattazione collettiva. Si tratta di norme immaginate per conseguire risparmi di risorse del bilancio dello Stato, in un momento storico-politico in cui l'andamento della spesa di risorse pubbliche è al centro dell'attenzione dell'Europa e dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Le mozioni trattano del rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine e delle Forze armate,

Sicuramente il tema del rinnovo dei contratti delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco non è nuovo al dibattito politico e questo Governo ha dimostrato attenzione al comparto già dallo scorso anno. Mi piace ricordare, infatti, il *bonus* previsto dalla legge di stabilità 2016 destinato al personale dei corpi di polizia, dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle capitanerie di porto: la gratifica di quasi 1.000 euro ha rappresentato un segno del riconoscimento dell'impegno di quegli uomini e quelle donne in divisa nel fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale. Inoltre se, come opportunamente ricordato dalla mozione a prima firma del senatore Gasparri, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale nel pubblico impiego, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, sottolineo che il disegno di legge di bilancio 2017 già individua le risorse necessarie per qualsiasi iniziativa di tipo negoziale. L'articolo 52 del disegno di legge, infatti, stanzia per il pubblico impiego quasi 2 miliardi di euro per il prossimo anno e oltre 2 miliardi e mezzo dal 2018. Tali risorse saranno destinate *in primis* ad incrementare i fondi già previsti a legislazione vigente con la legge di stabilità 2016 pari a 300 milioni di euro annui e finalizzati a finanziare i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Quindi, nell'ambito dei citati stanziamenti saranno individuati i soldi da destinare alle nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, compresi i corpi di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste necessarie a fronteggiare esigenze di servizio indifferibili e di particolare rilevanza ed urgenza. Infine, si prevede un incremento delle risorse previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale dei corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo dei vigili del fuoco, con l'obiettivo di attuare *in toto* la delega recata dalle norme della riforma della pubblica amministrazione.

come vediamo quotidianamente, affrontano rischi per tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone in un contesto ambientale e sociale estremamente turbolento, per cui meritano l'attenzione che il Parlamento dedica alla alla loro attività lavorativa, al loro impegno e spesso anche al loro sacrificio. Tale indicazione dà la cifra del percorso che si intende compiere e rappresenta l'elemento che farà da apripista ad ulteriori interventi di sostegno a settori del pubblico impiego, molto spesso trascurati dai soggetti che ne dovrebbero invece esaltare la specifica missione. Pertanto, il Gruppo di Area Popolare, coerentemente con gli impegni assunti in maggioranza e concretizzatisi nella manovra di bilancio, voterà a favore di tutti gli impegni volti a tutelare il grande operato dei Vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine e delle Forze armate per il nostro Paese.

cercando di trovare una soluzione; oppure, al contrario, il problema è risolto. Quindi, o è inutile il nostro lavoro, perché lei ha detto che è tutto a posto; o, al contrario, se il nostro lavoro è utile e impegna il Governo,

da parte di tutte le forze politiche per spingere il Governo a fare delle azioni, a fare qualcosa di concreto, posso solo supporre che quel «concreto» non c'è stato negli ultimi tre anni, altrimenti non ci sarebbe neanche bisogno di discutere di qualcosa che è già stato fatto da questo Governo. Evidentemente qualcosa non va. E io sono più convinto della seconda ipotesi, e cioè che lei sta dipingendo un quadro che non corrisponde alla realtà. Ma vale anche la prima ipotesi perché, malgrado il quadro non corrisponda alla realtà, neanche il nostro dibattito e il risultato delle mozioni e della loro votazione porteranno a qualche cambiamento, purtroppo. Lei ha espresso parere contrario ad alcune mozioni e parere favorevole ad altre. In particolare, lei ha espresso parere contrario a una mozione, a firma del Movimento 5 Stelle, che prevedeva di impegnare il Governo «ad incrementare significativamente ed in maniera strutturale le risorse economico-finanziarie destinate al comparto della sicurezza parere contrario «a prevedere il pieno ristoro del mancato adeguamento contrattuale dall'anno 2010 all'anno 2015»; parere contrario «a prevedere un piano straordinario di assunzioni nel settore della sicurezza e dell'ordine pubblico»; parere contrario assumere le opportune iniziative, di carattere normativo e regolamentare, affinché il personale (...) chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico sia munito, con assoluta urgenza, di sistemi idonei di equipaggiamento, con priorità per il personale operante in aree a rischio». Lei ha espresso parere contrario,

può che approvare. Io mi auguro che, malgrado il parere contrario, chi ha letto le mozioni si assuma la responsabilità di votare anche contro tutti i punti che ho testé elencato. Grazie a tutti.

facciamo dibattiti sulle interrogazioni dove sono presenti pochi parlamentari, e le interrogazioni sono un atto, se vogliamo, ancora più debole delle mozioni. Quindi, aver discusso delle mozioni è comunque utile, perché ci sono degli indirizzi. Sappiamo che essi indirizzi non sempre comportano decisioni cogenti e stringenti, né questo è il Parlamento: si fanno delle affermazioni e ciascuno di noi è chiamato - si ritiene - a risponderne. Che il dibattito sia stato utile - lo dico soprattutto al senatore Crimi, se

prima della legge di stabilità, mentre noi ci troviamo a discuterne l'8 novembre, con la legge di stabilità ancora *in itinere*. Mi illudo, ritengo e spero che anche il nostro atto di indirizzo parlamentare abbia

ai Gruppi parlamentari di proporre ulteriori stanziamenti. Almeno il mio Gruppo - lo so certamente - lo sta già facendo alla Camera, dove siamo in fase avanzata di discussione della legge di stabilità. Se la questione non si dovesse risolvere alla Camera, io lo farò al Senato.

Grazie a tutti.

Grazie a tutti. Quindi auguri a lei, Ministro, per le battaglie che dovrà condurre, perché i fondi dell'articolo 52 non bastano. Noi proporremo delle ulteriori misure. Come lei ha espresso parere favorevole alla nostra mozione, come è successo alla Camera, mi auguro che esprimerà parere favorevole anche sugli emendamenti che temo saranno necessari;

Grazie a tutti.

da questo Governo che ha invertito una tendenza e ha sicuramente operato per recuperare una situazione. Non abbiamo certo recuperato tutto quello che si è perso nel passato, ma abbiamo lavorato in un momento

Grazie a tutti.

un euro per la cultura, vuol dire che ci facciamo carico non solo di rispondere alle emergenze, ma anche di investire per il futuro del nostro Paese.

Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione. Passiamo alla

Presidente, la scorsa settimana a Genova un'intera famiglia è stata sterminata. Un uomo ha ucciso la moglie e le due figliolette prima di togliersi la vita. Apprendiamo che dietro questa tragedia si nascondevano grossi debiti causati dall'azzardo. Fuori dal clamore dell'attualità non possiamo dimenticarcene, perché questa volta non si trattava di *slot machine*. «Repubblica.it» sembra abbia pudore di parlare chiaro e dice asetticamente due volte «lotterie istantanee». Perché non si usa un termine che capiamo tutti? «Gratta e vinci»: gli innocui,

in cima alle preferenze dei ragazzi ci sono proprio i gratta e vinci. In secondo luogo, sono puntate a bassa latenza, e cioè passano pochi secondi tra l'acquisto e l'esito della puntata, e sappiamo, dunque, che hanno alto potere di dare dipendenza.

le combinazioni simili a quelle che farebbero vincere e che inducono a pensare - caspita - che si è vicini alla vittoria. Oppure le schede dispensano una miriade di microvincite per farci sentire bene e farci percepire che vincere sia facile, proprio come dice la pubblicità. Se ho puntato 5 euro e ricevo 5 euro, non ho vinto nulla, ma intanto mi viene dato un contentino. Si sa che così viene voglia di riprovarci e, puntualmente, il 95 per cento delle persone compra un nuovo biglietto e magari un altro ancora, perché la voglia rimane. dunque, di un'industria che studia la mente umana e i suoi meccanismi naturali, per torcerli contro le persone a vantaggio del *business* più spregiudicato. Non esiste un azzardo bonario i giornali lo devono dire chiaramente. Quando il sistema è concepito apposta per far male, non si può sostenere che a cascarci sono i deboli. Dovete accettare che l'azzardo è, di per sé, in grado di minare l'equilibrio delle persone. è dimostrato proprio da questo caso, perché l'autore del gesto disperato era un agente di polizia, una persona che i colleghi hanno definito equilibrata e che anche per lo Stato era capace di gestire un'arma al servizio dei cittadini. Dunque, mi chiedo chi sia veramente la mano omicida e quali responsabilità abbia un Governo che lascia dilagare questo commercio, senza nemmeno avere lo scrupolo di vietarne la pubblicità.

«Turista per sempre». Mi rivolgo al sottosegretario Baretta: sul divieto di pubblicità non ci può essere contropartita, è il minimo della decenza. Tutto il resto è scandalo.